Signor Presidente, l'istituzione di sezioni di liceo musicale rappresenta una delle più rilevanti innovazioni nel quadro della rivisitazione della formazione liceale con la inclusione, per la prima volta nella storia del nostro Paese, della musica tra i percorsi di base per la costruzione della persona di cultura. È palese che una svolta di questa rilevanza si rivela impegnativa dal momento che occorre assicurare fin dalla fase di decollo reali garanzie di qualità; da questo punto di vista, la collaborazione tra licei musicali e conservatori è uno degli assi per una concreta e funzionale strategia di

e, soprattutto, per una coerenza della nuova offerta formativa nell'ambito della domanda locale, delle tradizioni culturali e dei progetti di promozione della cultura musicale. È di tutta evidenza che il raggiungimento di intese richiede dialogo vero, reciproca fiducia, decisioni condivise e strategie comuni tra licei musicali e conservatori; a queste condizioni la realizzazione delle sezioni del liceo musicale può tradursi in una efficace azione diffusa che, nel medio periodo, può contribuire alla rivisitazione complessiva dell'intero impianto della formazione e della cultura musicale. Per quanto riguarda i criteri generali per l'individuazione dei nuovi licei musicali, che a parere dei senatori interroganti andrebbero rivisti, affinché le Regioni, nell'ambito delle proprie prerogative assumano gli atti conseguenti nei rispetto dei principi di equità e di uguaglianza, c'è da chiarire che essi già garantiscono quanto opportunamente richiesto nell'atto parlamentare. C'è infatti da sottolineare che, in via generale, sulla base di quanto disposto dal sopracitato sopracitato regolamento, inerente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, all'articolo 13, comma 6, le sezioni di liceo musicale e coreutica sono istituite nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Alla ripartizione delle sezioni a livello regionale si provvede comunque con riferimento ai criteri fissati in sede di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 64, comma

Per quanto riguarda la non attivazione di nuovo indirizzo del liceo di Sapri, richiesto in data 18 maggio all'assessorato istruzione della Giunta regionale della Campania e all'ufficio scolastico regionale della stessa Regione, si ritiene opportuno sottolineare, come riferito con nota n. 4200 della direzione generale per gli ordinamenti scolastici del MIUR e con nota n. 19746 dell'ufficio scolastico regionale competente, che la regione Campania non ha individuato il liceo «Pisacane» di Sapri quale destinatario dell'attivazione di un liceo musicale. L'istituto di Sapri non è stato infatti inserito, né nella delibera di giunta regionale n. 56 del 28 gennaio 2010 (avente oggetto: «Programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2010-2011») né nelle delibere successive di modifica e/o integrazione degli atti n. 201 del 5 marzo 2010 e n. 468 del 25 marzo 2010. L'inclusione nel piano di dimensionamento regionale è una delle condizioni fondamentali di avvio dei licei musicali, insieme al parere favorevole dell'ufficio scolastico regionale, all'esistenza documentata di strutture idonee, alla convenzione con un conservatorio di musica, alla disponibilità di risorse organiche e finanziarie. Si rappresenta, infine, che, in ogni caso, il liceo potrebbe proseguire il percorso di sperimentazione musicale intrapreso attraverso l'utilizzo della quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche con il DPR n. 89 del 2010 (articolo 10, comma 1, lettera *c)*).

può anche lasciare appagati, ma dal punto di vista politico restano in me tutte le perplessità che avevo manifestato durante il periodo precedente e che avevo cercato di esplicitare nell'interrogazione. Intanto, ringrazio lei ed il Governo per la risposta resa, ma chiedo un supplemento di impegno, e spiegherò perché. L'attivazione di un liceo musicale in un'area come quella del saprese, del Golfo di Policastro, che peraltro ella ben conosce, è semplicemente una modalità attraverso cui, come si addice ad una programmazione scolastica e ad una razionalizzazione della rete scolastica provinciale degne di questo nome, si possono assecondare una vocazione e una propensione a quel profilo formativo dei giovani del territorio anche coerente con un'antica tradizione - perché da qui deriva la domanda

poi un'altalena di pareri e di indicazioni: in una prima formulazione della Provincia di Salerno del 2009,

onorevole Sottosegretario, vi è piena coerenza con le indicazioni da lei stesso citate. Mi riferisco all'intesa con una istituzione musicale di carattere, tra l'altro, nazionale ‑ parlo del Conservatorio statale di musica «Martucci» di Salerno con cui da tempo il liceo «Carlo Pisacane» di Sapri ha stipulato una convenzione, un accordo di programma, tendente alla progettazione, al monitoraggio e alla valutazione di iniziative culturali relative all'educazione musicale, fin dal novembre 2009. 2009. Ci sono tutte le condizioni; tra l'altro, compare nel *curriculum*, nel corso degli anni, lo sviluppo di un percorso di sperimentazione musicale che si è concretizzato in numerosi progetti di educazione musicale, che non ripeto perché sono citati nella mia interrogazione.